sullo stato giuridico dei dipendenti pubblici e la riforma della dirigenza e su interventi di riordino di uffici e funzioni delle pubbliche amministrazioni, è in corso la diretta televisiva della RAI. Passiamo dunque alle interrogazioni sullo stato giuridico dei dipendenti pubblici e la riforma della dirigenza. I senatori hanno facoltà di rivolgere le loro domande al Ministro

A breve scadrà il termine entro il quale le varie istituzioni devono valutare la corrispondenza tra le funzioni e gli organici a disposizione, ad esempio per gli enti di area vasta.

ed agendo significativamente nel campo della durata degli incarichi dirigenziali. Tutto ciò, chiaramente, con l'idea di semplificare la pubblica amministrazione. Voglio concludere citando un altro elemento, che oggi anima la discussione che stiamo portando avanti in quest'Aula, ovvero il disegno

*(FI-PdL XVII)*. Signor Ministro, la tendenza del nostro ordinamento è sempre stata tesa ad equiparare la disciplina del lavoro pubblico a quella del lavoro privato. Ci chiediamo perché, dunque, stante l'assenza di qualsiasi norma contraria, il nuovo articolo 18 dello Statuto dei lavoratori riscritto dal *jobs act* non possa applicarsi agli oltre tre milioni di dipendenti pubblici presenti oggi in Italia. In merito alla riforma della dirigenza pubblica, vorrei poi richiamare l'attenzione del Ministro su un punto specifico: se vogliamo effettivamente riconoscere il merito, non si comprende per quale motivo la riforma diminuisca la parte della retribuzione legata al risultato, cioè quella con cui si premia chi concretamente raggiunge gli obiettivi. Una modifica proposta rinvia la definizione di tale quota al successivo decreto attuativo. Chiediamo, Ministro, perché la questione non sia definita subito, nell'ottica di valorizzare professionalità e merito dei dirigenti pubblici. Infine, la riforma della pubblica amministrazione prevede l'abolizione della carica di segretario comunale e provinciale. Proprio in questa figura la legge n. 190 del 2012 ha individuato il responsabile della prevenzione dei fenomeni corruttivi negli enti locali, mentre la riforma intende ora affidarsi solo alla figura del direttore generale, che costituisce l'emblema della mancanza d'imparzialità soggettiva, essendo di esclusiva scelta dei politici locali, che sono liberi di determinarne criteri di nomina e compensi. Le chiediamo, Ministro, se non sia più utile individuare una figura più autonoma, sul modello dei segretari comunali prima della riforma Bassanini. Signor Ministro, nelle amministrazioni statali abbiamo troppi dirigenti. Dovremmo, invece, ridurre i costi e, nello stesso tempo, promuovere il merito e le competenze. La separazione tra le prime e seconde aree di livello dirigenziale blocca ogni progressione verticale. All'area dirigenziale si accede da percorsi spesso estranei allo specifico contesto, frustrando le legittime aspirazioni dei funzionari che, ricordo, in molti casi sono laureati con *curriculum* di eccellenza, come nel caso del Ministero dell'economia e delle finanze, dove è richiesta la laurea con un punteggio minimo di 105. peraltro, porta a posizioni di delicata responsabilità persone che non hanno l'esperienza opportuna, spreca le risorse umane esistenti e quelle economiche, laddove si prevedono figure dirigenziali anche in strutture di minore complessità. Si chiede, pertanto, di conoscere la disponibilità a rivedere l'ordinamento del personale pubblico per ricostruire un percorso di sviluppo professionale, che una volta si chiamava carriera,

Si chiede, in particolare, se non sia il caso, proprio a tal fine, di istituire un'area di predirigenza con propria valenza giuridica, al fine di costituire posizioni intermedie tra dirigenti ed impiegati, dove collocare soggetti in grado di dirigere strutture di livello non necessariamente dirigenziale

compromesso dall'assenza di interventi tesi a ristabilire un riequilibrio tra il ruolo normativo della legge e il ruolo che spetta alla contrattazione collettiva, che negli anni, ahimè, è stato significativamente svuotato e ridotto a favore della prima, anche in relazione a materie collegate al rapporto di lavoro. Questa invasione di campo è avvenuta proprio in concomitanza di un fermo normativo della contrattazione collettiva, che si trascina ormai da quattro anni e che ha impedito, oltre gli adeguamenti retributivi, anche l'aggiornamento normativo dei contratti, i cui contenuti risultano ormai obsoleti rispetto ad un sistema economico e produttivo che negli ultimi anni ha subito una drammatica involuzione.

all'apertura della stagione contrattuale, anche per favorire quella profondità dell'intervento riformatore che ella stessa auspica per la pubblica amministrazione. Sulla questione della dirigenza, intervengo molto rapidamente. Non vorremmo che la concomitanza tra la legge delega e la disciplina per il personale delle Regioni e degli Enti locali, affidata all'articolo 11 del

per evitare che una lettura della norma in combinato disposto con quanto previsto dal decreto‑legge n. 90, ponga come criterio unico per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali il solo requisito fiduciario, prescindendo dal merito, dall'indipendenza nell'esercizio delle funzioni e da criteri di selezione trasparenti. Nutriamo dubbi sulla differenza dei due percorsi e non vorremmo che la severità proposta per la regolazione della dirigenza di merito servisse poi a far entrare nella pubblica amministrazione

È di questa settimana una trasmissione televisiva abbastanza goliardica che ha citato il caso di un unico dirigente di un comune che attribuisce tutto il premio della produttività al segretario generale:

quale sia l'approccio della riforma della pubblica amministrazione che proprio in questi giorni stiamo discutendo in Commissione affari costituzionali in Senato.

sia davvero fondamentale per migliorare la democrazia del nostro Paese, perché laddove i servizi pubblici vengono erogati in modo semplice e trasparente ci troviamo in un

essere una risposta anche per tutte quelle lavoratrici e per quei lavoratori pubblici che in questi anni si sono sentiti travolti da una rappresentazione decadente dell'amministrazione che non li rispecchia, perché ogni giorno lavorano con

di chi oggi lavora nell'amministrazione pubblica, sia importante proprio nella direzione del merito. Nella riforma della pubblica amministrazione puntiamo su una dirigenza

tolto le percentuali rigide sull'indennità di risultato perché pensiamo che addirittura la carriera del dirigente debba essere legata alla valutazione e al merito. Pensiamo che il merito e la valutazione debbano

una parte importante della discussione parlamentare, e quindi della riforma, proprio su meccanismi che, garantendo l'autonomia e l'indipendenza della dirigenza, ne garantiscano anche

cancellando le attuali funzioni dei segretari comunali: con una fase transitoria, stiamo piuttosto attribuendo queste funzioni fondamentali ad un dirigente di ruolo autonomo ed indipendente dalla politica, quindi non chiamato

manteniamo lo scarso rendimento come ragione del procedimento disciplinare e, semplificandolo, facciamo in modo che chi non fa bene

che il dipendente sia proprietà privata di una singola amministrazione. L'amministrazione è un corpo unico, è la Repubblica del nostro Paese.

infatti, devono stare per il tempo giusto nel posto giusto, laddove servono a fornire un servizio alla collettività. Ogni dipendente è dipendente della Repubblica e credo che questa sia la migliore risposta alla valorizzazione di quel lavoratore che, prima di tutto, vuole essere inserito in un'organizzazione del lavoro che gli consenta di essere un servitore dello Stato, un servitore della Repubblica. Credo davvero che questa riforma, anche per altri aspetti che non ho tempo di discutere

L'organizzazione dello Stato, della pubblica amministrazione deve essere strutturata in modo tale da rendere difficile, e comunque complicato, poter accedere

C'è stata un'ampia condivisione nell'abolizione, tra tre anni, della figura del segretario comunale; figura intesa come indispensabile per garantire lo svolgimento delle funzioni locali in autonomia e nel rispetto della legalità e a garanzia non tanto degli amministratori quanto dei cittadini. E qui risalta proprio la funzione amministrativa rispetto a quella politica. Infatti, la garanzia che l'imparzialità sia realizzata grava sull'apparato amministrativo. In questo senso, la figura del direttore generale, generale, uno dei principali fallimenti delle riforme Bassanini, configura invece una situazione di equilibrio precario perché posizionata tra politica e burocrazia, ognuna con le sue logiche, spesso in contrasto. Questo vale anche per la prevenzione dei fenomeni di corruzione negli enti locali.

Lei ha parlato dell'amministrazione come di un corpo unico, ma a me sembra che voi vogliate trapiantare su un corpo che ha una sua organicità una testa estranea, con dirigenti che magari non hanno alcuna esperienza di quello specifico settore. Si parla di mobilità orizzontale anziché parlare della progressione verticale ed è lì dove possiamo valorizzare il merito. Quanto all'ipotesi di istituire una predirigenza, anche ai fini di ridurre i costi, lei non ha risposto, ma immagino che su questo ci confronteremo in Commissione. Credo

ma dando la possibilità di accedere a funzioni più complesse e più gratificanti, perché è questo che sta demotivando i nostri dipendenti pubblici e i funzionari. sulla riapertura della stagione contrattuale lei è qui a dirci che ce ne sono le condizioni, se la riforma andrà

MANASSERO *(PD)*. Signor Ministro, come lei ha appena ricordato nella premessa della sua risposta, siamo nel pieno di un percorso di riforme: quelle dello Stato, delle autonomie, dei rapporti con le Regioni e della pubblica amministrazione all'interno di questo quadro, intendo sottoporre a lei, signor Ministro, ed al Governo la questione del presidio del territorio. Abbiamo un bisogno urgente di riforme, siamo stati troppo fermi ed oggi ne sentiamo tutto il peso e ne paghiamo l'intero prezzo, ma abbiamo bisogno di buone norme che ci restituiscano uno Stato ed una pubblica amministrazione efficienti e moderni, più vicini ai cittadini ed in grado di garantire maggiore democrazia. In questo quadro, provo ad elencare alcune delle priorità rispetto alle quali è indispensabile mantenere un attento presidio di legalità e presenza sui nostri territori: territori: le amministrazioni locali, i nostri Comuni, i sindaci ed i tantissimi amministratori. Il lavoro puntuale della Commissione di inchiesta sulle intimidazioni rivolte agli amministratori locali che è stato svolto da questa Camera ci racconta delle loro difficoltà: sono soggetti a pressioni ed azioni di ricatto ed intimidazione, fenomeno che fa fatica ad emergere chiaramente ma che esiste, lo leggiamo negli atti e nelle cronache e mina il rapporto tra cittadini e politica. È quindi necessario riorganizzare la presenza periferica dello Stato per rompere la solitudine degli amministratori. poi i fenomeni corruttivi legati agli appalti e alle nomine, e il bisogno di semplificare i procedimenti e l'organizzazione delle strutture, ma senza venir meno alla garanzia della legalità degli atti e della loro efficacia. Penso in questo caso alla presenza di figure nei Comuni e in tutti quei soggetti che devono spendere denaro pubblico per investire e fornire servizi ai nostri concittadini. *(FI-PdL XVII)*. Signor Ministro, il progetto di riforma della pubblica amministrazione prevede la riorganizzazione degli apparati pubblici statali, intervenendo su Ministeri, agenzie governative, forze di polizia e prefetture. Questa razionalizzazione dovrebbe consentire di risparmiare soldi pubblici, da destinare ai servizi ai cittadini. Tuttavia, per poter valutare la riforma di quella che è stata definita la più grande azienda del Paese, ci sono questioni che vanno necessariamente chiarite. Le chiediamo quindi se la riduzione delle forze di polizia colpirà il solo Corpo forestale e in che modo, nel merito, il Governo intenda procedere in questa operazione di assorbimento, e quali altre forze di polizia saranno coinvolte. Chiediamo se se sia stato fatto un censimento di quanti, pur facendo parte delle forze dell'ordine, sono impiegati in lavori d'ufficio anziché di controllo dell'ordine pubblico infine, a che punto sia arrivato il procedimento per ricollocare quei 20.000 dipendenti delle Province in esubero che continuano ad attendere dal Governo soluzioni d'impiego alternative. C'è infatti il rischio concreto che il processo di mobilità del personale venga slegato dal trasferimento delle funzioni, al contrario di quanto previsto dalla legge n. 56 del 2014. un significativo numero di dipendenti provinciali in sovrannumero potrebbe transitare verso Regioni, Comuni e amministrazioni statali per svolgere mansioni totalmente diverse da quelle precedenti. Signora Ministra, l'articolo 7 del disegno di legge n. 1577 contiene una delega concernente la riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato. la lucidità del disegno governativo, mirante soprattutto alla riduzione degli apparati pubblici, è messa in dubbio dalla stessa Corte dei conti, che riscontra l'esigenza di un coordinamento con la normativa vigente e di considerare gli effetti delle riforme già avviate nella stessa direzione. La Corte, tra l'altro, osserva: «A fronte di un più ampio orizzonte di riforma, quale emerge dalla stessa finalità della previsione di delega, intesa a privilegiare il ruolo di servizio della pubblica amministrazione ai cittadini ed alle imprese, un obiettivo da perseguire è quello di una rivisitazione delle dimensioni, del ruolo e delle attribuzioni degli uffici, da attuare attraverso un percorso di razionalizzazione degli apparati in stretta aderenza alle funzioni perseguite e non solo in termini quantitativi». Più precisamente, «tale percorso di razionalizzazione richiede una attenta verifica delle funzioni svolte, anche alla luce di un possibile ripensamento del complessivo perimetro di intervento, a fronte delle competenze demandate ai livelli territoriali e ad altri soggetti pubblici». Sicché, «in questa logica di fondo, in cui pare muoversi anche il disegno di legge all'esame, potrebbero rendersi maggiormente espliciti gli ambiti di definizione della delega». Insomma, la Corte si permette di ricordare al Governo il fondamentale insegnamento di Massimo Severo Giannini, secondo cui «in principio sono le funzioni», e cioè il principio in base al quale i problemi relativi all'organizzazione, al personale, alle procedure di una pubblica amministrazione sono conseguenti e quindi accessori a quello principale relativo alle funzioni della medesima amministrazione. A tal proposito, chiediamo al Ministro quali siano i numeri relativi a razionalizzazione e riorganizzazione dei pubblici uffici, considerando il criterio funzionalistico e necessario degli stessi, che il Governo ha calcolato unitamente ai risparmi che tutto ciò dovrebbe portare alla spesa pubblica ed ai conti dello Stato. In un'ottica di funzionalismo riconosciuto della pubblica amministrazione, si domanda poi se il Ministro intenda perseguire un'attività

*(Misto-ILC)*. Signor Ministro, ci stiamo apprestando a riformare la pubblica amministrazione con il disegno di legge che avete presentato Un aspetto che viene all'evidenza dell'utenza, dei cittadini che si rivolgono alla pubblica amministrazione, è che spesso, a fronte di sforzi da parte degli impiegati che vi lavorano, i servizi non sono adeguati alla richiesta. Abbiamo rilevato che l'attività di programmazione annuale della pubblica amministrazione presenta alcune criticità, la prima delle quali è che spesso il programma non viene definito prima che sia trascorsa la metà dell'anno cui fa riferimento. L'altra criticità è che spesso gli obiettivi, che a quel programma sono parametrati, sono al di sotto della capacità operativa della struttura amministrativa, cioè quest'ultima non è spinta dal soggetto politico a operare al massimo delle sue capacità. Chiediamo quindi al Governo se è disponibile a far partecipare i cittadini, tramite associazioni di utenti, all'attività di programmazione, a far apprezzare il programma così definito ed il livello di conseguimento degli obiettivi che spesso, come abbiamo visto, è attestato dagli stessi dirigenti che quegli obiettivi dovrebbero aver conseguito.

nella vostra volontà di modificare il funzionamento dell'attività amministrativa.

oggi si è operato con pratiche spesso contrarie al principio di buona amministrazione. In larga parte, questo è stato anche imputabile all'assenza di criteri e procedure di valutazione in grado di misurare l'efficienza dell'operato delle diverse pubbliche amministrazioni, rilevando scostamenti rispetto alla gestione *standard* o alle gestioni più virtuose. La legge n. 42 del 2009, infatti, aveva previsto il superamento del tradizionale criterio della spesa storica e l'introduzione di percorsi obbligati di reimpostazione delle politiche della pubblica amministrazione sulla base dei costi *standard*. Del resto, questi avrebbero potuto offrire un contributo alla prevenzione dei fenomeni di corruzione. Secondo noi, sarebbe opportuno, anche al fine di razionalizzare i costi, introdurre un sistema di articolazione della spesa pubblica basato sull'individuazione dei fabbisogni

tutti gli interventi di riforma, dall'attuazione della legge Delrio, che supera il livello di governo delle Province, al disegno di legge Boschi di riforma del Titolo V della le ragioni innumerevoli di conflitti di attribuzione che ci sono stati in questi anni tra Stato e Regioni, fino all'articolo 7 della delega che stiamo discutendo in Commissioni affari costituzionali qui in Senato e che é il cuore della riforma della pubblica amministrazione, hanno

un unico ufficio territoriale che rappresenti lo Stato e il Governo per i cittadini e che, quindi, eviti che il cittadino quando deve

per affermare il principio che l'amministrazione è una, che non è una sommatoria di amministrazioni e che, in quanto corpo unico, rappresenta la Repubblica e quindi lo Stato per quel cittadino che ha il diritto di ricevere servizi pubblici con tempi e regole certe. Tutti gli interventi quindi sono volti a razionalizzare, a cancellare le duplicazioni e a semplificare per

e alla gestione, per esempio, di tutte le pratiche legali o del personale. Nelle forze di polizia vogliamo superare le duplicazioni

ricollocare le competenze che oggi non servono più alle Provincia per svolgere le funzioni essenziali - così come le definisce la legge Delrio - fra tutte le altre amministrazioni. Subito dopo la legge di stabilità, abbiamo emanato una circolare che chiarisce come deve essere attuata su questo punto la legge di stabilità; stiamo ultimando e ci accingiamo a presentare le tabelle di equiparazione che devono servire a capire come queste persone vengono inquadrate e quindi all'inquadramento quale quale retribuzione corrisponda, con la cautela che non ci siano perdite retributive; stiamo per emanare un decreto che contiene i criteri per la mobilità Regione per Regione; partecipiamo ad incontri quotidiani, anche informali,

realizzando la più grande operazione di mobilità che ci sia mai stata nella storia repubblicana. Le cose le stiamo facendo e su questo vi chiedo veramente aiuto e collaborazione, affinché sempre meglio e sempre più velocemente queste persone possano svolgere una funzione che che valorizzi le loro competenze nel posto giusto, per il tempo giusto e dove quelle competenze servono, appunto, a fornire un servizio al cittadino. Per quanto riguarda il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini, senatore Endrizzi, ne abbiamo fatto una regola sempre e comunque. L'agenda per la semplificazione - composta da 38 azioni che stiamo monitorando nella loro attuazione, con un cronoprogramma dettagliato, che dura tre anni - è frutto

che si possa anche solo avvicinare a un taglio lineare, ma allo stesso tempo vogliamo evitare qualunque tipo di inefficienza e di spreco, abbiamo scelto di fare della trasparenza un'azione profonda profonda e costante del Governo. Abbiamo promosso un sito Internet, che abbiamo chiamato soldipubblici.gov.it, che vogliamo migliorare, rendendolo all'altezza delle migliori pratiche inglesi e statunitensi. Vogliamo che, laddove ci sono risorse

e di accompagnamento, soprattutto per quanto riguarda il mondo dei lavoratori, che naturalmente non sono scoperti, ma vanno in qualche modo guidati e accompagnati.

e che la sua circolare sul personale delle Province ha tentato di mettere una pezza sulla situazione, oggettivamente insostenibile, determinata dalla riforma, dal momento che l'unica disposizione pienamente attuata della riforma Delrio è stato il cambio alla guida degli organi politici.

una compressione della pubblica amministrazione operando tagli lineari. Ma, di fatto, in passato sono stati fatti solo e soltanto tagli lineari. Quando si parla di blocco del*turnover*, ad esempio, si fa riferimento all'intera pubblica amministrazione. Ora, fermo restando che questi sono certamente lasciti di precedenti Esecutivi, si era chiesto semplicemente se era stata avviata una severa e rigorosa indagine per capire dove si annidassero disfunzionalità. È certamente auspicabile che il sito che lei ha indicato - soldipubblici.gov.it - dia uno strumento al cittadino per capire come e cosa si sia fatto e si possa fare, ma è altrettanto vero che alle parole dobbiamo far seguire i fatti. pertanto, che vi siano indicazioni più precise, perché siamo convinti che la spesa pubblica, relativamente al funzionamento della pubblica amministrazione, non sia eccessiva o esagerata, ma sia, piuttosto, mal distribuita.

nella preparazione della riforma della pubblica amministrazione, sia nella preparazione di "buona scuola", chiedendo quali fossero i *desiderata* dei cittadini. Io non parlavo di quello, ma di cosa serve ai cittadini, nel concreto, nel programma di un anno e di cosa pensano i cittadini - controllo successivo - dell'attività dell'amministrazione con cui vengono in contatto, che è altro rispetto a una serie di richieste molto vaghe su un aspetto amplissimo: nessuno cittadino può controllare l'effettiva rispondenza tra quanto chiede e quanto poi il Governo dà, così come sta avvenendo. Tant'è vero che, ad esempio, a livello di buona scuola, ma ma anche nella pubblica amministrazione, il nostro timore è che il risultato finale sarà assai distante e distinto dalle richieste dei cittadini.

Si chiama *question time*: *question*, domande. Noi veniamo a porre domande dirette e lei ci risponde elencando le linee guida del Governo sulla riforma della pubblica amministrazione. Questa cosa va benissimo, ma la deve fare in Commissione: va lì e spiega. In questa sede lei ci deve solo dare delle risposte. Ho parlato di costi *standard* Ho sentito parlare della riforma della polizia: tutte cose cui nessun collega in quest'Aula ha accennato. Ci viene anche a prendere in giro, due volte, quando ci dice «vogliamo uno Stato più semplice e più snello». Significherebbe uno Stato dimagrito, significherebbe andare verso una riforma federalista. Lei usa anche terminologie centraliste: la Repubblica, lo Stato, la pubblica amministrazione. Ma la riforma delle pubbliche amministrazioni l'avete fatta togliendo alle Regioni quelle poche competenze che avevano: tutte le competenze complementari e secondarie delle Regioni adesso sono in capo allo Stato; demolite e togliete competenze anche alle Regioni e alle Province a statuto speciale. Sul fronte dei Comuni avete raggiunto il massimo di tagli di tagli agli enti locali: nemmeno Monti o Letta avevano fatto i tagli drastici operati dal vostro Governo. Ma come potete venire con faccia angelica a prendere in giro il Senato? Al *question time* non ha dato una risposta a nessuno. La propaganda la dovete fare con altri strumenti, in altri luoghi, adattissimi: questo non è il luogo per fare propaganda politica. Qui il suo ruolo è dare risposte a domande che non avremo altra occasione o altro modo di formulare in modo diretto.